mi è parso che il senatore Segretario abbia detto che mancava il parere della Commissione finanze. Non voglio attribuire al presidente

Il decreto-legge fu discusso e approvato da una maggioranza anche più ampia di quella tradizionale; poi è stato emanato il decreto attuativo,

quale alla fine dell’anno terminerebbe - uso il condizionale, naturalmente - il quantitative easing. Questo rende ancor più serio e drammatico il problema,

convocazione PRESIDENTE. Informo che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni, che costituisce l’unico punto all’ordine del giorno della seduta antimeridiana odierna. Pertanto, Pertanto, il seguito della discussione del provvedimento proseguirà in altra seduta, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo. Comunico inoltre che nella seduta pomeridiana di martedì 30 maggio, alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori.

Con lettera in data odierna i senatori Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di Giacomo, Fucksia, Giovanardi e Quagliariello hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI), indicando quale Presidente del Gruppo il senatore Quagliariello, Vice Presidenti le senatrici Bonfrisco e Fucksia e Tesoriere il senatore Davico. Pertanto i senatori Augello, Compagna, Davico, Giovanardi e Quagliariello cessano di appartenere al Gruppo GAL, le senatrici Bonfrisco e Fucksia cessano di appartenere al Gruppo Misto, il senatore Aracri cessa di appartenere al Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, i senatori Bilardi e Di Giacomo

Signora Presidente, come ha giustamente rilevato la collega Comaroli - evidentemente oggi è la giornata in cui le opposizioni prendono le difese della Commissione bilancio il problema è non solo e non tanto che non è responsabilità della Commissione bilancio non avere adempiuto all’obbligo di fornire il parere di merito sulla legge che riguarda i diritti delle persone sorde e sordocieche. Il problema, piuttosto, è un altro: non si può continuare a pensare di legiferare con leggi manifesto che non hanno necessaria e sufficiente copertura, come evidenziato dagli interventi dei membri del Gruppo di Forza Italia durante il dibattito. Questo è un problema oggettivo, perché il mancato riscontro ed il mancato contributo da parte della Ragioneria generale dello Stato di ciò che serve per mandare avanti questa norma è legata al fatto che, onestamente, in questa circostanza si sono evocati diritti senza avere la capacità

intervengo solo per rassicurare i colleghi e per spiegare almeno in parte il motivo di questo ritardo. Il tema, paradossalmente, non è la copertura finanziaria, come ricordava il senatore Mario Mauro, anzi il ritardo è legato al fatto che

fortunatamente si è scoperto che molte delle previsioni inserite come norma quadro in questo provvedimento ricevevano già una copertura finanziaria da altra normativa esistente. abbiamo limato la capienza finanziaria di questo provvedimento e quindi resta semplicemente di avere contezza del risultato finale.

lo ha testimoniato con le parole di molti colleghi) di mettere al centro per la prima volta il tema della comunità sorda nel nostro Paese e di offrire una visione complessiva anche rispetto ai diversi orientamenti

per la manovrina che impegna il Ministero alla Camera, lo dobbiamo dire con molta franchezza. Spero che in questo fine settimana le cose si sistemino,